Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prefettura di Catania ha riferito che presso l'Ufficio scolastico provinciale di quella città opera, già da alcuni anni, un gruppo di lavoro composto da docenti con lo specifico compito di svolgere un'attività di monitoraggio volta esclusivamente a volta esclusivamente a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. L'attività del predetto gruppo di lavoro ha portato alla realizzazione di una rete interistituzionale composta da 41 Osservatori integrati d'area che coprono l'intero territorio provinciale. Il gruppo effettua un monitoraggio degli alunni a rischio dispersione, analizzandone le cause ed intraprendendo azioni finalizzate a risolvere le problematiche emerse: tali iniziative, attuate spesso in sinergia con l'Ufficio provinciale del lavoro, talvolta richiedono - per poter essere efficaci - il trattamento di dati sensibili, per il quale i docenti sono stati regolarmente e formalmente autorizzati. Il predetto gruppo anti-dispersione, durante il corrente anno scolastico, oltre alla consueta rilevazione dei dati ha focalizzato l'attenzione sugli studenti stranieri e sulle loro difficoltà di integrazione, sulla base di quanto emerso dagli incontri con i coordinatori di alcuni Osservatori d'area nei cui ambiti territoriali nei cui ambiti territoriali insistono insediamenti nomadi, ma anche tenendo presente il protocollo d'intesa per la tutela dei minori rom, sinti e camminanti stipulato in data 24 aprile 2009 tra il MIUR e l'Opera nomadi. Per dare attuazione all'iniziativa il gruppo ha inviato alle scuole della Provincia una scheda di rilevazione la cui finalità era quella di «porre in essere eventuali interventi a favore degli alunni immigrati che in atto frequentano le istituzioni scolastiche di questa Provincia», recando l'avvertenza che, trattandosi di dati sensibili, la scheda doveva essere consegnata *brevi manu* al personale autorizzato. Faccio presente che i dati acquisiti sono stati utilizzati anche per elaborare strategie di intervento per la partecipazione ad un bando FEI (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi) al quale lo stesso Ufficio ha aderito, in qualità di *partner*, con un progetto interistituzionale insieme alla Provincia regionale di Catania (ente capofila) e con il coinvolgimento anche dell'Università degli studi di Catania e di un ente operante nell'ambito del sociale. La prefettura di Catania, considerata la rilevanza sociale dell'iniziativa, si è limitata esclusivamente a segnalare la pubblicazione del bando FEI agli enti pubblici interessati, ma non ha in alcun modo partecipato alla raccolta dei dati, né tanto meno alla conservazione degli stessi. Tali dati, infatti, non sono stati trasmessi ad alcun ente esterno e rimarranno custoditi presso l'Ufficio scolastico provinciale, per essere trattati al solo scopo di porre in essere iniziative volte a combattere la dispersione scolastica in favore degli alunni extracomunitari che attualmente frequentano le istituzioni scolastiche della Provincia.

L'interrogazione era nata soprattutto a seguito di un articolo apparso su «l'Unità», che parlava di schedatura di tutti i cittadini stranieri, a seguito di una nota della prefettura presso tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Catania. Era piuttosto singolare che questa iniziativa riguardasse solo la città di Catania e non le altre Province siciliane. Per tale ragione avevamo firmato questa interrogazione, cioè per chiedere

Il Sottosegretario ci parla di un'iniziativa della prefettura di Catania nell'ambito di un progetto per la dispersione scolastica. Faccio notare che questi progetti del MIUR riguardano tutte le scuole italiane:

non posso che stigmatizzare l'atteggiamento delle istituzioni scolastiche di Catania, che hanno inteso con questa iniziativa, peraltro abbastanza arbitraria, non solo schedare gli immigrati irregolari, ma soprattutto utilizzarne dati sensibili, cosa peraltro proibita dalla legge. Questa volta debbo dire che sono soddisfatta della risposta, perché conferma la denuncia presente nell'articolo apparso su «l'Unità» il 3 febbraio 2010. Spero che non si possano ripetere casi del genere, perché tutte le scuole sono impegnate nel progetto contro la dispersione scolastica;

che mai possono essere utilizzati. Spero che il Ministero possa, a questo punto, controllare come vengono utilizzati tali dati e verificare perché il provveditorato di Catania abbia inteso raccoglierli. Spero anche che episodi del genere non possano più ripetersi in